Premesso che: si susseguono quotidianamente scambi polemici tra il Presidente del Consiglio dei ministri Renzi e le istituzioni dell'Unione europea; è sempre più forte l'impressione che manchi al Governo italiano una strategia forte e che difetti la capacità di perseguire un chiaro e serio disegno europeo, a fronte di una situazione economica oggettivamente compromessa e di una propensione a spinte antieuropeiste crescente nel Paese. nel Paese. La politica non può abdicare al suo ruolo, lasciando spazio ad impulsi e paure collettive o, peggio, scivolando nel populismo; la querula insistenza da parte del Governo italiano presso la Commissione europea per ottenere ulteriore flessibilità sembra mostrare una debolezza intrinseca e un respiro corto, molto simile alle richieste avanzate dal quarto Governo Berlusconi nel 2011. Si tratta di una politica che mira solo ad ottenere vantaggi nazionali, che spesso vengono utilizzati in chiave elettoralistica (penso agli 80 euro e alla cancellazione della Probabilmente occorrerebbe incalzare l'Europa al rispetto, da parte della Commissione, dell'impegno preso per una politica di crescita degli investimenti, con grandi progetti comuni che possano fare da volano, creando nel contempo margini di ulteriore flessibilità condivisa sui bilanci. Il cosiddetto partito dell'austerità si combatte creando un fronte riformista contrapposto ai conservatori, allargando le intese europee per decisioni condivise su grandi temi come l'immigrazione e la crescita. La risposta non può essere un ripiegamento puro e semplice sulla difesa delle politiche nazionali, rivendicando maggior spazio per le politiche di bilancio nazionali, ma il dispiegarsi di una vasta azione aggregatrice e di conquista del consenso per fare un balzo in avanti nell'integrazione: affiancare ai molti fattori, già oggi integrati in Europa, quello più importante e non ancora integrato, la politica, che, attraverso scelte nuove e coraggiose, può far superare visioni anguste e restrittive, come l'austerità e le politiche recessive di bilancio. La via maestra per affermare questa visione di ampio respiro non può che consistere nel sollecitare progetti di investimento a livello europeo, finanziati con risorse del bilancio dell'Unione, ovvero facendo ricorso al mercato per opere straordinarie (pensiamo alla situazione del

sarebbe importante puntare ad una proposta rivolta all'insieme dei Paesi dell'area euro, soprattutto in quei Paesi in cui si manifestano particolari esigenze di maggiore integrazione. Per questo vorremmo sapere dal Presidente del Consiglio dei ministri se non ritenga necessario informare il Parlamento sulla situazione attuale in Europa

Informiamo regolarmente, nella persona del Presidente del Consiglio, il Parlamento sulle scelte di politica europea dell'Italia prima di ogni Consiglio europeo; lo facciamo dopo, attraverso la presenza del sottoscritto e di altri membri del Governo; diamo informazioni sistematiche attraverso numerosissime audizioni dei vari membri del Governo in materia di politica europea; trasmettiamo in maniera puntuale le relazioni programmatiche e consuntive di politica europea del Governo e diamo una comunicazione puntuale su tutte le procedure di infrazione infrazione richieste dal Parlamento. Quindi non credo, obiettivamente, che, se qualcosa manca, questa sia l'informazione. Il Parlamento è pienamente informato della politica europea del Governo e ha ampiamente occasione Il secondo aspetto che oggi ha sollevato - ce ne sono altri nell'interpellanza - è il tema dei Trattati. non abbiamo mai fatto mistero di voler sfruttare innanzitutto tutti gli strumenti esistenti nei Trattati europei per andare verso lo sviluppo di politiche nell'interesse dell'Italia e dell'Europa su temi che sono prioritari per quanto riguarda l'agenda italiana e l'agenda europea: la politica dell'immigrazione, la politica della sicurezza e la politica economica. Su questo abbiamo da tempo superato il tabù e la paura di parlare di revisione dei trattati. Se si realizzassero

non solo una piena attuazione dei trattati da leggere alla luce delle nuove priorità, ma anche una revisione dei trattati (un tabù che il Governo Renzi ha superato da vario tempo), saremo certamente pronti a fare la nostra parte. Noi però non vogliamo aspettare; vogliamo lavorare per creare un vero dibattito transnazionale e sviluppare le politiche europee, ovviamente alla luce delle scelte del Governo Renzi, ma nell'interesse di un avanzamento dell'integrazione politica di tutta l'Europa. È per questo che, d'intesa con le tre Presidenze di turno attuali (olandese, slovacca nel secondo semestre di quest'anno e maltese nel primo semestre del prossimo anno), abbiamo avviato un dibattito transnazionale che si svolge in vari Stati membri, con la partecipazione di membri del Parlamento

di una vera, nuova fase di integrazione politica, che deve vedere nella politica di crescita, di lotta contro la disoccupazione, di immigrazione e dei diritti fondamentali dello Stato di diritto, i tre pilastri del rilancio. Da ultimo, lei, nell'interpellanza e in particolare nell'intervento di oggi, invitato il Governo a svolgere un'azione volta all'uscita dalle fallimentari politiche di austerità. Se c'è un Governo che negli ultimi due anni ha con forza rimesso in questione le politiche dell'austerità, e con forza, ma senza rotture, con la forza delle idee, delle riforme e della politica, portato avanti una visione alternativa delle politiche economiche della zona euro, questo - me lo lasci dire - è proprio il Governo italiano. E la stessa flessibilità, che ha avuto un momento importante proprio ieri - le raccomandazioni rivolte all'Italia oltre che ad altri Paesi della Commissione europea non fanno altro che confermare la strategia del Governo italiano - non è un'eccezione fatta all'Italia, ma un'applicazione a tutta la zona euro, in maniera più intelligente, cioè più favorevole alla crescita, all'occupazione e agli investimenti, delle regole comuni. Quindi è un lavoro che noi abbiamo fatto sulla base di scelte nazionali, ma di cui beneficia, con questo approccio molto più aperto, l'intera zona euro e che ci sembra avere avuto ieri un altro momento di dialogo positivo. Non vedo tensioni fra noi e la Commissione europea, come lei ha evocato oggi. Siamo entrati in una fase di dialogo molto costruttivo e credo che la decisione di ieri ieri relativa alla legge di stabilità italiana, le proposte della Commissione europea sulla revisione delle regole di Dublino e sulla creazione di un corpo di polizia europeo delle frontiere esterne, l'accoglienza molto positiva da parte della Commissione europea e di altri Governi dell'Unione europea della proposta italiana in materia di immigrazione e di rapporti tra Europa ed Africa (*immigration compact*), che ha una componente di investimenti e sviluppo e una componente di cooperazione in materia di immigrazione,

onorevole Sottosegretario, la ringrazio per la sua cortesia. Non sono soddisfatto della risposta poiché, a fronte di una serie di dichiarazioni che effettivamente ricalcano quanto lei ha detto, c'è un discorso di sostanza. Mi spiego.

vengono definiti periferici rispetto all'Unione. Penso alla Grecia: ricordo quando si è ritrovata nella trattativa tra Tsipras e la Commissione, tra Tsipras e i Paesi del Centro Europa. Sarebbe stato auspicabile da parte dell'Italia un un atteggiamento di maggiore solidarietà, che sicuramente sarebbe stato utile sia alla Grecia che all'Italia Per quanto riguarda la possibilità di una maggiore elasticità nell'impiego del bilancio e la disponibilità di 14 miliardi in più, rilevo che, per gli impegni assunti contestualmente dal nostro Governo,

dagli interroganti, vorrei precisare alcuni aspetti relativi innanzitutto al ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Dipartimento per le politiche europee che svolge compiti di coordinamento e di monitoraggio in materia di aiuti di Stato, ivi inclusa la predisposizione di relazioni trimestrali sulle procedure di indagine formali e sui recuperi, mentre sono le singole amministrazioni pubbliche - che si tratti di Ministeri, di Regioni o enti locali - ad essere responsabili per gli aiuti concessi e gli eventuali recuperi. Al fine di consentire alle autorità concedenti gli aiuti l'acquisizione delle informazioni e dei dati concernenti la lista dei soggetti destinatari degli aiuti incompatibili che devono restituire e anche per evitare ai medesimi l'erogazione di nuovi aiuti, il Dipartimento per le politiche europee ha predisposto e pubblicato sul suo sito l'elenco delle decisioni che dispongono il recupero degli aiuti di Stato individuali. Sono ben lieto di rispondere a future interpellanze per informazioni più generali. Vi invito regolarmente, anche ogni giorno se volete, a consultare il sito che abbiamo predisposto. Inoltre, per quanto riguarda l'elenco delle imprese interessate dalle decisioni che dispongono il recupero del regime degli aiuti di Stato, il Dipartimento per le politiche europee lo ha reso accessibile, previa domanda delle amministrazioni concedenti aiuti di Stato da formulare agli indirizzi PEC delle singole amministrazioni che curano i recuperi degli aiuti. I medesimi sono sempre pubblicati sul medesimo sito di cui sopra dal 31 dicembre 2015. I dati contenuti in elenco che consente di verificare in sede istruttoria per la concessione di nuovi aiuti la posizione dei beneficiari che devono restituire gli aiuti illegali e incompatibili - confluiranno in un nuovo Registro nazionale degli aiuti che sarà operativo dal gennaio 2017. Con riferimento, in maniera specifica, ai casi che avete citato, vorrei segnalare che le amministrazioni competenti, sempre in conformità alla normativa europea e alla legge n. n. 234 del 2012, hanno posto in essere tutte le azioni necessarie per i recuperi. L'esistenza dei casi per i quali non si è potuto dare corso alle procedure esecutive con carattere di immediatezza è dovuta alla presenza di molteplici contenziosi pendenti nei diversi gradi di giudizio. Di seguito si forniscono, quindi, le informazioni relative alle misure adottate dalle singole amministrazioni per il recupero di aiuti di Stato illegali e incompatibili per le quali la Commissione europea ha ordinato il recupero, con propria decisione. Vorrei sottolineare che l'esatta quantificazione delle somme che devono considerarsi recuperate è, comunque, sempre - è la disciplina degli aiuti di Stato soggetta alla valutazione finale della Commissione europea. Pertanto, i dati forniti di seguito non possono considerarsi definitivi prima di un riscontro formale ricevuto dalla Commissione europea.

Il primo tema è relativo agli sgravi fiscali alle imprese site a Venezia e a Chioggia. L'importo complessivo dovuto alle aziende alla data del 1° marzo 2016 è stato quantificato in 36.353.832,93 a titolo di sorte capitale e in 67.113.253,62 euro quali interessi in misura composta. Per quanto concerne la sorte capitale sono stati recuperati circa 20 milioni di euro. Per quanto riguarda la misura relativa agli interessi da applicare (tasso semplice o composto) il Consiglio di Stato si è riservato ogni decisione in merito, rinviando a successiva udienza, per la quale non è tuttavia ancora intervenuto il provvedimento di fissazione. di fissazione. Si resta quindi in attesa di tale pronuncia, per conoscere la misura esatta degli interessi da applicare. Il secondo caso che gli interroganti hanno sollevato è il cosiddetto caso Occupazione Pacchetto Treu. Alla data del 1° marzo 2016, tenuto conto anche delle valutazioni rese nella nostra interlocuzione con la Commissione europea in ordine ai progressi che abbiamo svolto, come Italia, nell'attività di recupero, le aziende considerate sanzionabili sono 158, con un importo da recuperare (sorte capitale) pari a 40.414.769,49 di euro, rispetto agli originari circa 331 milioni di euro. Anche in tal caso, la non immediata esecuzione deriva dalla mancata definizione dei ricorsi pendenti in Cassazione. Il terzo caso riguarda le aziende ex municipalizzate. municipalizzate. L'importo complessivo soggetto a recupero è di circa 770 milioni di euro di sorte capitale. In data 27 febbraio 2012, a fronte delle ingenti somme recuperate, la Commissione europea ha sospeso formalmente la decisione di deferire l'Italia alla Corte di giustizia ai sensi dell'articolo 260 del Trattato di funzionamento dell'Unione europea. Alla data del 27 aprile 2016, l'importo ancora da recuperare è di 1.877.451,12 a titolo di capitale, oltre gli interessi comunitari da rideterminare alla data di effettivo pagamento. Ne consegue che, a tale data, è stato recuperato il 99,6 per cento dell'aiuto inizialmente da recuperare. Sui recuperi residui pende un contenzioso in ordine al tipo di interesse da applicare (semplice o composto). Pertanto, si resta in attesa delle relative pronunce, per conoscere la misura degli interessi da applicare. quarto caso riguarda Euroallumina. La società Eurallumina sta procedendo alla restituzione degli aiuti ricevuti, ancorché in misura parziale. I dati dovranno essere forniti dall'Agenzia delle dogane, competente al recupero. La società medesima ha prodotto due ricorsi innanzi al TAR Sardegna per l'annullamento, previa sospensiva degli atti di revoca di rateizzazione e di intimazione al pagamento. L'udienza per l'esame del ricorso sulla sospensione è fissata per il 13 luglio 2016. Il quinto caso è relativo alla proroga della legge Tremonti-*bis*. Il procedimento di recupero ha riguardato sia coloro che hanno fruito dell'aiuto in conformità alla legge nazionale cosiddetta "beneficiari", sia i soggetti che hanno beneficiato della misura agevolativa in violazione della stessa normativa interna cosiddetta "evasori". Relativamente ai "beneficiari", il recupero è stato ultimato nel 2014. Rispetto ai soggetti "evasori", alla data del 27 aprile 2016, ad avviso delle autorità competenti al recupero, sono stati riscossi e definiti procedimenti per circa 20 milioni di euro ed attualmente sono in corso procedure di riscossione coattiva nei confronti di 4 posizioni residue

Il recupero riguarda il settore alberghiero e, alla data del 21 aprile 2016, risulta in corso. Esso viene effettuato, in stretto raccordo con la Commissione europea, secondo un piano di recupero con pagamenti da effettuare entro ottobre 2016. Hanno concretamente aderito a tale piano di pagamento nove imprese. Per alcune di quelle che non hanno aderito al piano di recupero è stata avviata la procedura esecutiva. Una impresa è stata pignorata, ed un'altra è stata dichiarata fallita. Il settimo caso è quello della Sardinia Ferries: l'importo dell'aiuto da recuperare in questo caso ammonta a 2,1 milioni di euro (sorte capitale). I soggetti tenuti alla restituzione dell'aiuto sono due, rispettivamente per il 90 e per il 10 per cento. Entrambi i beneficiari hanno instaurato un contenzioso sul recupero. A seguito del rigetto delle loro richieste, in data 7 febbraio 2016, Equitalia, incaricata della riscossione coattiva, ha avviato le procedure esecutive. In data 24 marzo 2016,

L'ottavo caso concerne la SACE BT: gli aiuti da recuperare riguardano due ricapitalizzazioni a SACE BT, rispettivamente per 29 e 41 milioni di euro. In esecuzione degli obblighi di recupero, è stato emanato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 16003 del 3 agosto 2015, volto al recupero delle misure di aiuto di Stato. Al riguardo, SACE BT SpA ha comunicato informazioni volte, tra l'altro, a dimostrare l'avvenuto recupero degli aiuti di Stato. Il nono caso è quello della Sea Handling: La Commissione europea nel qualificare il complesso dei conferimenti effettuati da Sea SpA a Sea Handling come aiuto di Stato illegale ed incompatibile con il mercato interno, ha ordinato all'Italia il recupero dell'aiuto, per un ammontare di 359,644 milioni di capitale. Ai fini del recupero, considerato che la concessione dell'aiuto viene indiscutibilmente imputata al Comune di Milano, quest'ultimo è l'autorità nazionale che deve adottare le procedure amministrative necessarie per assicurare l'esecuzione della decisione. Avverso tale decisione, Sea Handling e il Comune di Milano hanno presentato ricorso - tuttora pendente - presso il competente tribunale europeo. Nelle more del recupero è stata avviata la procedura di liquidazione della società Sea Handling e la costituzione di un nuovo soggetto (Airport Handling). La Commissione europea il 9 luglio 2014 ha adottato una decisione di avvio di indagine formale, nella quale ha sollevato il dubbio che la liquidazione di Sea Handling e la contestuale creazione di Airport Handling possano costituire una mancata esecuzione della propria decisione di recupero del 2012. La decisione definitiva, che dovrà essere adottata dalla Commissione europea, chiarirà se Airport Handling è in rapporto di discontinuità economica con Sea Handling ormai posta in liquidazione - in qual caso, ovviamente, non si parlerebbe di aiuti di Stato - e quindi se l'obbligo di restituzione gravante su Sea Handling si sia trasferito o meno su Airport Handling. Questo dipende ovviamente dalla valutazione sulla discontinuità economica che la Commissione europea darà, alla luce delle informazioni ricevute. Il decimo caso riguarda Saremar: la decisione della Commissione ha riguardato la compensazione per oneri di servizio pubblico erogata (10 milioni di euro) e la ricapitalizzazione di Saremar (824.309,60 euro). In data 1° luglio 2014 Saremar SpA ha presentato ricorso per concordato preventivo volto a consentire la dismissione dell'intero complesso aziendale ed il soddisfacimento con il ricavato dei terzi creditori. La procedura concordataria ha previsto la vendita degli *asset* da parte dei liquidatori giudiziali, che si è conclusa con l'aggiudicazione della flotta navale. Effettuata la vendita del naviglio e la fine delle attività di cabotaggio, il curatore dovrà riunire il comitato dei creditori ed indicare l'importo che potrà essere realmente recuperato, per poi procedere alla liquidazione. L'undicesimo e penultimo caso, Presidente, sollevato dagli interroganti, concerne CSTP e Buonotourist, entrambi di competenza della Regione Campania. In attuazione della decisione della Commissione europea del 19 novembre 2015, in data 18 marzo 2016, Campania, competente per il recupero, ha ingiunto alla società CSTP di restituire l'importo relativo all'aiuto di Stato illegale. A seguito del mancato pagamento nei termini, è stato attivato il procedimento per la riscossione coattiva tramite Equitalia, che ha notificato la cartella esattoriale. La Buonotourist Srl ha fatto ricorso innanzi al TAR Campania, che ha disposto l'interruzione della procedura di riscossione coattiva.

Gli ultimi due casi sono relativi alle agevolazioni fiscali e contributive in Abruzzo e ai vantaggi fiscali per compensare i danni del terremoto in Sicilia e altre calamità naturali. Con la decisione del 14 agosto 2015, riguardante i casi di aiuti di Stato SA.33083 e SA.35083, relativi alle agevolazioni tributarie, previdenziali e assicurative

ha chiesto di effettuare il completo recupero degli aiuti concessi a seguito del sisma che ha colpito l'Abruzzo nel 2009, ma solamente per le agevolazioni in sovracompensazione dei danni e per importi superiori a 200.000 euro. Con riferimento agli altri eventi calamitosi risalenti nel tempo, il recupero riguarda solo le imprese, ove esistenti, che hanno beneficiato dell'aiuto pur avendo solo sede legale e non operativa Le operazioni finalizzate al recupero rientrano nelle competenze del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L'ammontare degli importi da recuperare sarà determinato a seguito delle operazioni di elaborazione dei dati relativi alle tre tipologie di benefici concessi per ogni beneficiario nella sola misura

Nella mia interrogazione ho citato dei casi che partono dal 1999, passando per il 2004, fino al 2014. Le dico, per inciso, che a tutt'oggi abbiamo la bellezza di 62 casi di procedura di infrazione per violazione del diritto dell'Unione

abbiamo pagato una penalità di 65.280 euro (sembra niente, ma la cifra è per ogni giorno di ritardo) e la bellezza di 7.140 euro (sempre al giorno) per il periodo intercorso tra la sentenza del 2006 e la seconda sentenza della Corte questo per avere un'idea di quanto ci costano i mancati adempimenti. Eppure, già nel 2007 la Commissione aveva comunicato quali fossero le migliori pratiche volte a garantire una più rapida e integrale esecuzione delle decisioni,

rispetti le norme sugli aiuti di Stato. Poiché è in corso una gara, voglio avvisare i vari Arvedi, Marcegaglia, i turchi di Erdemir e soprattutto i cittadini italiani, visto che dentro c'è Cassa depositi e prestiti,

Signor Presidente, signor sottosegretario Gozi, avevo preparato un intervento per il tempo che mi era stato assegnato, ma ritengo che il collega Castaldi abbia ben sintetizzato la nostra posizione.

Credo che noi non dovremmo neanche arrivare a queste sanzioni e a questi contenziosi. Inoltre vediamo che solo alcune società ben note usufruiscono di aiuti di Stato, che poi magari - come

come noto, numerose sono le iniziative e gli interventi voluti dal Ministro della Giustizia per innovare il sistema carcerario nella sua complessità, in un'ottica che si propone di rimeditare il concetto di esecuzione della pena, con l'obiettivo di conferire adeguate condizioni di dignità e vivibilità non soltanto ai ristretti, ma anche agli operatori. Infatti, sono stati emanati decreti ministeriali di chiusura di alcuni istituti con caratteristiche non più adeguate al nuovo modello detentivo ed è, altresì, proseguita l'attività istituzionale volta alla riqualificazione e alla valorizzazione del patrimonio demaniale in uso governativo all'amministrazione penitenziaria. Inoltre, in seguito alla chiusura anticipata al 31 luglio 2014 del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie, è stato riattivato il Comitato paritetico interministeriale per l'edilizia penitenziaria, costituto da rappresentanti del Ministero della giustizia e del Dicastero delle infrastrutture e dei trasporti, con il proposito di avviare un programma di modifica del piano carceri, per aggiornarlo al mutato quadro di fabbisogni territoriali rispetto alla situazione delineata nel 2009 e al diverso modello di detenzione che si intende attivare. Deve essere evidenziato che, in questo contesto, la competente Amministrazione ha già provveduto a verificare le condizioni strutturali della casa di reclusione di Padova e ad attivarsi per adottare le soluzioni più opportune. Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha riferito, al riguardo, che, a seguito del sopralluogo effettuato alla fine del mese di ottobre dello scorso anno dal personale tecnico, il locale provveditorato ha richiesto l'assegnazione di una somma pari a 1.500.000 euro, per provvedere ad un intervento di ripristino delle finiture edilizie e degli impianti. Compatibilmente con le risorse assegnate è intendimento dell'Amministrazione penitenziaria provvedere ad inserire, nell'ambito della programmazione degli interventi dei prossimi esercizi finanziari, lavori di manutenzione straordinaria di carattere generale, mirati al ripristino della piena funzionalità del penitenziario padovano, nei quali sarebbe ricompresa anche la caserma annessa all'istituto. La caserma annessa alla Casa di reclusione di Padova è una palazzina di dieci piani, con 160 camere da tre e da due posti, aventi una metratura di 37 e 33 metri quadri ciascuna e da camere singole, con adeguati servizi esclusivi. Le camere sono tutte abitabili, dotate di bagno ed idonee allo scopo cui vengono adibite. Con riferimento alla previsione del pagamento di un canone per alcune unità abitative, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha riferito che si tratta di un mero contributo per le utenze, pari per la camera singola a 37,35 euro mensili, per la camera doppia a 64,17 euro mensili e per camera tripla a 70,13 euro mensili. La predetta Amministrazione ha altresì precisato che, in ossequio alla direttiva del Ministro della giustizia 31 ottobre 2013, adottata ai sensi dell'articolo 17, lettera *d)*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è stata operata una distinzione fra camere di pernottamento delle caserme agenti ed alloggi ad uso collettivo *ex* articolo 12, n. 314 del 2006. Per le prime non è previsto l'obbligo di versamento di alcun canone, in quanto «strutture rispondenti a finalità di prevalente interesse istituzionale, poiché strumentali a favorire la permanenza del personale presso gli istituti medesimi e che non possono essere riservate a un determinato occupante fuori dei giorni di effettivo utilizzo». Per gli altri alloggi, invece, trattandosi di un utilizzo esclusivo degli spazi collettivi di servizio, è stato individuato, a carico degli occupanti, un canone di concessione pari ad una quota forfettaria giornaliera commisurata ai soli servizi o consumi. Tali unità abitative possono, dunque, essere assegnate in via esclusiva al personale che faccia richiesta di averle per un uso personale e continuativo, dietro la corresponsione di una quota forfettaria, che rappresenta il corrispettivo dei servizi connessi al normale uso dell'alloggio. Resta comunque fermo il possibile utilizzo delle stesse a titolo gratuito, ove ricorrano esigenze istituzionali e di servizio.

nell'autunno successivo si sono mossi i primi interventi, ma le ristrutturazioni partiranno solo nei prossimi esercizi finanziari. Vi è una situazione gravissima: la polizia penitenziaria, che ha un ruolo delicato, è proprio delicato, è proprio stremata. Devono garantire la sicurezza dei cittadini, ma anche dei detenuti; devono usare la forza e rispettare la dignità della persona e, in questo compito, si trovano drammaticamente sotto organico, mentre i detenuti sono in condizioni di sovraffollamento. In base agli ultimi dati, in Germania ogni 100 posti ci sono 82 detenuti, in Spagna 85, in Inghilterra 97. In Italia ogni 100 posti abbiamo 108 detenuti, ma i dati sono falsati

E se è indegno che i detenuti siano ammassati in strutture fatiscenti, pur avendo responsabilità penali da scontare, è inaccettabile che siano destinati alloggi fatiscenti a chi in queste strutture svolge un servizio per la Nazione. Nell'interrogazione che ho presentato la situazione del carcere «Due Palazzi» è emblematica, peraltro, di una condizione sistemica. Gli agenti di polizia penitenziaria vengono ospitati - si fa per dire, visto che devono anche pagare - in strutture totalmente inadeguate, con la conseguenza che alcuni, molti, scelgono di provvedere autonomamente, con disagi evidenti che non sono solo di natura economica, perché la retribuzione non copre senz'altro la responsabilità, i rischi e le pressioni sopportate, ma dovendo spostarsi anche lontano, visto che il carcere è fuori dalle zone residenziali, aumentano i disagi di spostamento e non è una questione meramente privata o personale. Il pronto intervento degli agenti, in situazioni di emergenza, deve essere considerato una priorità. La possibilità di soggiornare presso le strutture non può essere considerata un privilegio ma uno strumento a servizio dell'interesse collettivo e per il Ministero dovrebbe rappresentare una responsabilità etica, un elemento di credibilità politica. A pochi chilometri da Padova, emerge poi la vicenda scandalosa del nuovo penitenziario di Rovigo, costato 29 milioni di euro e di fatto non funzionante. Non funzionano la caserma, gli alloggi, la mensa per gli agenti, mancano del tutto i servizi come spaccio, sale ricreative e palestra e tra Padova e Rovigo gli agenti penitenziari sono sotto organico del 50 per cento e quindi sono costretti a turni massacranti, a volte in condizioni igienico-sanitarie non sempre ottimali. Altro caso è il carcere di Vicenza, dove pochi mesi fa i sindacati di polizia penitenziaria hanno denunciato la presenza di vermi nei piatti serviti alla mensa. Anche qui, di fronte ad una capienza di 156 posti, i detenuti erano 216 con il padiglione destinato ai collaboratori di giustizia sovraffollato del doppio rispetto all'effettiva capacità. Ricordo che il Movimento 5 Stelle aveva presentato tre anni or sono un piano carceri, con un costo nettamente inferiore rispetto al programma del Governo che si trova ora a doverlo rettificare. Avrebbe peraltro consentito di risolvere il problema del sovraffollamento senza ricorrere ad amnistie, indulti o sanatorie che offendono il senso di giustizia dei cittadini. Come spesso accade, siamo rimasti inascoltati ed oggi la situazione che vive la polizia penitenziaria è questa: alloggi fatiscenti, turni massacranti, straordinari non pagati e aggressioni subite, perché il numero di detenuti è sproporzionato rispetto a quello degli agenti. Allora, vede, sulla vicenda del carcere di Padova non è accettabile che il Governo si sgravi la coscienza dicendo che in fin dei conti pagano poco perché stiamo parlando di alloggi che, comunque, non sono abitazioni (non hanno la possibilità di ospitare nemmeno un amico o di ricevere una visita), sono alloggi strettamente di servizio e allora, a questo punto, devono essere anche totalmente gratuiti e dignitosi. Invito il Governo il Governo a valutare la situazione senza avere il timore di ammettere il fallimento. È un dovere che lo Stato ha nei confronti dei cittadini onesti e che pagano le tasse e chiedo un sollecito intervento, netto ed urgente, per sopperire al malfunzionamento del carcere di Padova e delle altre strutture penitenziarie venete.

Ha infatti introdotto il principio per cui nelle liste dei candidati al consiglio comunale è assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi. Nelle medesime liste, nei Comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi. Analogamente, con riferimento all'elezione dei Consigli comunali nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, «nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi». Queste disposizioni sono volte a promuovere la parità di uomini e donne nell'accesso alle cariche elettive, attraverso un prestabilito bilanciamento delle candidature di entrambi i sessi nelle elezioni amministrative che riguardano i Comuni con popolazione non inferiore a 5.000 abitanti. Dal tenore letterale delle disposizioni si evince con estrema chiarezza che le soglie massima dei due terzi e minima di un terzo, nell'eventualità in cui il correlato numero contenga una cifra decimale, sono comunque determinate mediante l'applicazione del criterio dell'arrotondamento matematico. A titolo esemplificativo, nell'ipotesi in cui il numero massimo dei candidati di una lista corrisponda a 16 (nei Comuni con abitanti al di sopra dei 10.000 e al di sotto dei 15.000), 15.000), essendo i due terzi pari a 10,66 ed un terzo pari a 5,33, sulla base del criterio il risultato porterebbe al riparto delle candidature in rappresentanza dei due sessi nei limiti massimo e minimo, rispettivamente, di 11 e 5. La Direzione centrale dei servizi elettorali del Ministero dell'interno ha inizialmente fatto propria tale interpretazione letterale della norma nella circolare n. 30 del 2013. A partire dal mese di settembre 2014, ha invece improvvisamente modificato il suo orientamento, per aver il Governo accolto un ordine del giorno della Camera dei deputati, precisamente il 31 luglio del 31 luglio 2014, nella parte in cui lo impegnava "a modificare, conformemente alla volontà espressa dal legislatore nel corso dei lavori volta a favorire al massimo la rappresentanza di genere, l'interpretazione fornita nella circolare n.30/2013, applicando nella formazione delle liste elettorali il criterio dell'arrotondamento all'unità superiore, anziché il criterio dell'arrotondamento aritmetico"; tale mutamento di indirizzo è stato subito recepito nella circolare ministeriale n. 37 del 13 settembre 2014 e reso noto ai sindaci ed ai presidenti delle commissioni e sottocommissioni elettorali attraverso apposite comunicazioni prefettizie, peraltro, il testo delle richiamate norme è talmente chiaro da non lasciare spazio a dubbi interpretativi di sorta. E non è un caso che lo stesso Ministero abbia, nella fase iniziale, correttamente aderito ad un'interpretazione letterale, per poi ribaltarla solo in accoglimento dell'ordine del giorno; tali rilievi sono confermati

contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi" preclude in radice la possibilità di sostenere l'applicabilità del criterio dell'arrotondamento all'unità superiore, dovendo trovare applicazione il criterio di arrotondamento aritmetico, il quale, peraltro, ha sempre costituito il parametro il principio in base al quale l'interpretazione della legge è operazione che deve essere condotta secondo criteri fissati con priorità, pertanto, del criterio dell'interpretazione letterale; ciò con la conseguenza che l'interpretazione da prescegliere non può essere che quella che risulti il più possibile aderente al senso letterale delle parole,

alcuna valenza può essere riconnessa né alle istruzioni per la presentazione e per l'ammissione delle candidature, né alla circolare del Ministero dell'Interno n. 37 del 16 settembre 2014, risultando all'evidenza ostativi i fondamentali principi in materia di gerarchia delle fonti; come correttamente rilevato dalla difesa di parte ricorrente, infatti, la circostanza che il Governo abbia accolto un ordine del giorno discusso dalla Camera dei Deputati dei Deputati nel luglio 2014 con l'impegno a "modificare l'interpretazione ....applicando nella formazione delle liste elettorali il criterio dell'arrotondamento all'unità superiore, anziché il criterio (...) aritmetico" non è, di per sé, sufficiente a determinare alcuna efficacia innovativa nell'ordinamento, risultando all'uopo necessaria una modifica della formulazione della disposizione in esame"»; sono ormai imminenti le elezioni comunali ed è necessario chiarire la questione, anche al fine di scongiurare incertezze e contenziosi, signor sottosegretario Bocci, le chiediamo di chiarire definitivamente i dubbi interpretativi finora emersi, riaffermando la piena e letterale applicazione dell'articolo 2, comma 1, della legge 23 novembre 2012, n. 215, che ha introdotto le modifiche agli articoli 71 e 73 del testo unico per gli enti locali.

si chiedono chiarimenti definitivi in merito all'interpretazione delle disposizioni introdotte con la legge n. 215 del 2012, che regolano il riparto delle candidature in rappresentanza dei due sessi nella formazione delle liste elettorali. Gli interpellanti ritengono che tali disposizioni abbiano accolto, per il calcolo della cosiddetta quota rosa, il criterio dell'arrotondamento aritmetico, cioè dell'arrotondamento all'unità più vicina, e a conforto del loro orientamento richiamano la sentenza, così come è stato ricordato, del TAR Campania n. 2589 del 2015. Invero, come ricordato nell'interpellanza, in un primo tempo il Ministero dell'interno, Direzione centrale dei servizi elettorali, aveva emanato la circolare esplicativa n. 30 del 2013, ispirata proprio al criterio dell'arrotondamento aritmetico. Successivamente, tuttavia, il Governo, come ha ricordato nell'illustrazione, ha accolto un ordine del giorno della Camera dei deputati, esattamente del 31 luglio 2014, impegnandosi a dare applicazione al diverso criterio, che è quello, com'è stato sottolineato, dell'arrotondamento all'unità superiore, conformemente alla volontà espressa dal legislatore nel corso dei lavori parlamentari, volta a favorire la massima rappresentanza di genere. Di conseguenza, questa amministrazione si è attivata per recepire il nuovo orientamento e ha diramato la circolare n. 37 del 13 settembre 2014 anch'essa citata nell'interpellanza - con la quale sono state fornite specifiche indicazioni in ordine all'ammissione delle liste elettorali in linea con il nuovo criterio di calcolo delle quote della rappresentanza di genere. In particolare, è stato esplicitato che l'arrotondamento all'unità superiore riguarda, anche in caso di cifra decimale inferiore a 50 centesimi, il numero minimo, com'è noto, pari a un terzo dei candidati del genere meno numeroso in ciascuna lista nelle elezioni dei Comuni con almeno 5.000 abitanti. modalità di arrotondamento trovano applicazione sia nei Comuni con popolazione compresa tra i 5.000 e 15.000 abitanti, sia in quelli con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, ferme restando le rispettive modalità di ripristino del rapporto tra i generi in lista, dì competenza delle commissioni e sottocommissioni elettorali, previste dalla legge. Tanto detto e passando a rispondere al quesito contenuto nell'atto di sindacato ispettivo, ritengo che, in presenza del succitato impegno del Governo, questa amministrazione potrà considerare l'opportunità di cambiare l'attuale indirizzo nel senso auspicato dai senatori interpellanti, e cioè nel senso di adottare il diverso criterio dell'arrotondamento all'unità più vicina, qualora si formi e si consolidi, in seno al Consiglio di Stato, un conforme orientamento giurisprudenziale.

su questa materia la funzionalità democratica dei consigli comunali, anche in ossequio alle cosiddette quote rosa, ha una priorità assoluta. Pertanto, nel ribadire il mio

senatori, il senatore Caridi, nel sottolineare l'importanza della prefettura di Vibo Valentia, quale presidio di legalità in una provincia densa di problemi sotto il profilo della sicurezza pubblica e dell'immigrazione, chiede di soprassedere alla sua chiusura, prevista da uno schema di regolamento governativo di riorganizzazione delle strutture centrali e territoriali del Ministero dell'interno. Il tema evidenziato è particolarmente sentito nell'opinione pubblica locale, che ha dato vita a una forte mobilitazione sfociata nell'autunno dello scorso anno in una manifestazione alla quale hanno preso parte cittadini, amministratori locali ed esponenti del mondo sindacale, associativo e produttivo di quella Provincia. Anche il Consiglio regionale della Calabria si è occupato del problema, approvando all'unanimità una mozione contro il taglio dei presidi statali nel territorio vibonese. Al riguardo, faccio subito rilevare che lo schema di regolamento in questione appartiene a una stagione di rigore sotto il profilo economico-finanziario, sancita nel decreto-legge n. 95 del 2012, in cui la *spending review* faceva premio su tutto il resto dei bisogni e delle esigenze. Ora però la direzione imboccata è un'altra. Non che le esigenze di contenimento della spesa pubblica siano venute meno, ma il Governo ha accolto l'idea che la razionalizzazione della presenza dello Stato sul territorio debba debba essere ispirata, da un lato, a criteri di sostenibilità sociale e, dall'altro, debba accompagnarsi alla valorizzazione del ruolo delle prefetture. Questo cambio di rotta lo troviamo suggellato nella cosiddetta legge Madia, che pur prefigurando la riduzione del numero delle prefetture, sulla base di una serie di indicatori oggettivi legati all'andamento della criminalità, all'esposizione ai flussi migratori e alle dinamiche socioeconomiche nei territori di competenza, ne rafforza la funzione strategica. Ciò è attestato dal fatto che esse andranno ad assorbire tutti gli uffici periferici dello Stato e si configureranno, quindi, quali punti di contatto unico tra lo Stato e i cittadini. Le prefetture, inoltre, continueranno ad essere il cardine del sistema territoriale della sicurezza. Va segnalato peraltro che, in base a una disposizione della legge di stabilità 2016, il regolamento governativo su cui vertono le due interrogazioni all'ordine del giorno dovrà essere adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo dei criteri di delega della cosiddetta In sostanza, solo dopo l'approvazione - non ancora intervenuta - di quest'ultimo decreto sarà possibile mettere mano in concreto al regolamento sulle prefetture, tenendo conto di tutte le argomentazioni esposte in precedenza. Al momento, quindi, nessuna prefettura sarà accorpata. Sui contenuti del regolamento per la loro riorganizzazione, vi sarà anche lo spazio per un confronto serio e approfondito con le istituzioni locali, che tenga conto delle istanze provenienti dal territorio. Assicuro fin d'ora che l'attuale articolazione periferica del Ministero dell'interno, costituita dalle prefetture, dalle questure e dalle strutture periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, non risulterà modificata dal nuovo disegno ordinamentale, in coerenza con il modello di unitarietà territoriale delle autorità di pubblica sicurezza e delle Forze di polizia di cui alla legge n. 121 del 1981, con effetti favorevoli sulla presenza dei presidi di sicurezza sul territorio. In una delle due interrogazioni si chiede anche quali azioni si intendano porre in essere affinché siano rafforzati i presidi di sicurezza e di tutte le Forze di polizia presenti nella provincia di Vibo Valentia. Al riguardo, rappresento che il dispositivo delle Forze dell'ordine dispiegato in quel territorio si compone complessivamente di 1.424 unità. In tale ambito, gli appartenenti ai ruoli operativi della Polizia di Stato sono 406, rispetto ad una previsione organica di 297 unità, con un sovrannumero di 109 operatori, ai quali si aggiungono 18 appartenenti ai ruoli tecnici. Sono presenti, inoltre, 608 militari dell'Arma dei carabinieri e 392 militari della Guardia di finanza. Le dotazioni dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza appena citate sono state incrementate di recente e costituiscono, al momento, il massimo sforzo organizzativo possibile per i due corpi di polizia, tenuto conto degli analoghi impegni di pubblica sicurezza su tutto il territorio nazionale. Aggiungo che, al fine di ottimizzare l'impiego degli organici territoriali, i servizi di prevenzione generale vengono, di volta in volta, rimodulati nel corso di apposite riunioni tecniche interforze, sulla base di criticità riscontrate e secondo specifiche strategie che garantiscono sempre un'adeguata presenza di operatori delle Forze dell'ordine Inoltre, in occasione di servizi straordinari di prevenzione generale, il dispositivo territoriale di polizia viene supportato da aliquote regionali dei reparti prevenzione crimine della Polizia di Stato e delle compagnie di di intervento operativo dell'Arma dei carabinieri. mi tranquillizza l'aumento delle Forze dell'ordine per presidiare un territorio difficile come quello di Vibo Valentia e, in generale, calabrese. Nel caso della prefettura di Vibo Valentia, ho voluto mettere in evidenza la difficoltà dei tanti sindaci e amministratori e delle tante imprese che giornalmente lavorano su quel territorio. Mi tranquillizza anche il fatto che lei dica che al momento la prefettura di Vibo Valentia non sarà chiusa, ma voglio questa garanzia anche per il futuro. Non si si può parlare di soppressione, anzi bisogna rafforzare quei territori che necessitano di sicurezza per dare tranquillità agli operatori economici e soprattutto, ai cittadini.

Signor Presidente, con l'interrogazione all'ordine del giorno la senatrice Gambaro, unitamente ad altri, pone l'attenzione sul *deficit* di rappresentanza che si sarebbe venuto a determinare nelle comunità degli *ex* Comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio e Savigno per effetto della loro fusione nel nuovo Comune di Valsamoggia. Premetto che la riunificazione di questi Comuni del bolognese è avvenuta nel solco di una normativa statale e regionale che da tempo incentiva la creazione di percorsi di unificazione tra Comuni, al fine di realizzare la semplificazione e razionalizzazione dei servizi con effetti positivi non solo sulle finanze pubbliche ma soprattutto sugli investimenti nei territori di competenza. II legislatore ha peraltro tenuto presente come tale tipo di operazione porti con sé il rischio di un affievolimento dell'identità territoriale, prevedendo, proprio per evitare tale evenienza, modalità di coinvolgimento e partecipazione delle comunità che vanno a fondersi. Desidero anche ricordare che la fusione dei cinque Comuni costituisce il risultato di un percorso di aggregazione culturale e umana, avviato da anni dalle comunità dei Comuni citati e di altri limitrofi, che avevano già dato luogo all'unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia. Il Comune di Valsamoggia è stato istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, con la legge regionale n. 1 del 2013, che ha demandato allo statuto l'eventuale istituzione dei municipi nei territori delle comunità di origine o di alcune di esse. Cogliendo tale opportunità, lo statuto comunale di Valsamoggia ha previsto l'istituzione dei municipi, quali organi di partecipazione che rappresentano ì territori delle comunità di origine, ne curano gli interessi, ne promuovono lo sviluppo nell'ambito dell'unitarietà del Comune in questione e si impegnano a tutelare i diritti individuali delle persone, l'ambiente e il territorio di competenza. è stato previsto che nei territori degli *ex* Comuni, accanto agli organi del Comune nuovo, ossia sindaco, Giunta e Consiglio comunale, operino i municipi con funzioni di iniziativa, proposta, consulenza e vigilanza sullo svolgimento dei servizi e delle attività comunali di interesse delle predette comunità. Organi di ciascuno dei cinque municipi sono il consiglio di municipio e il presidente. Il consiglio è composto da dieci persone elette a suffragio diretto con sistema proporzionale, contestualmente al Consiglio comunale. Tenuto conto che i municipi sono cinque, il numero complessivo dei consiglieri è di 50. Tanto detto, quanto alle dimissioni cui fanno riferimento gli interroganti, evidenzio che esse sono state rassegnate da 17 dei 18 consiglieri di municipio di minoranza, appartenenti alla Lista Civicamente Samoggia. A seguito delle dimissioni, i cinque consigli di municipio, espletati i procedimenti di surroga, hanno preso atto, con proprie deliberazioni, della rinuncia alla nomina di consigliere di municipio da parte di tutti i candidati della citata lista, tranne a Savigno, dove si è verificata la surroga di un consigliere dimissionario. Il Comune di Valsamoggia ha comunicato, che, a conclusione delle vicende istituzionali appena descritte, i consigli municipali continuano ad avere una composizione numerica tale da consentire il regolare funzionamento di tali istituzioni e la salvaguardia della rappresentanza delle singole comunità locali. Infatti, in ogni municipio è presente un numero di consiglieri superiore alla metà degli stessi, in linea con quanto previsto dal regolamento dei municipi, in vigore dal 14 agosto 2014, secondo cui il consiglio di municipio si riunisce validamente quando è presente almeno la metà dei consiglieri assegnati. In ordine, invece, all'esigenza di una più dettagliata e specifica disciplina normativa in tema di fusione di Comuni, finalizzata a salvaguardare le istanze delle singole comunità, rilevo che, a seguito della modifica intervenuta con la cosiddetta legge Delrio (la legge n. 2014), è stato ulteriormente specificato che lo statuto del Comune risultante da fusione «può prevedere anche forme particolari di collegamento tra nuovo Comune e comunità appartenenti ai Comuni fusi». Il Parlamento ha quindi riservato all'autonomia dei singoli enti locali - con esclusione di spazi di intervento statuale - l'individuazione delle modalità attraverso le quali salvaguardare i profili di identità e di partecipazione in quelle realtà che, in attuazione di una razionalizzazione abbiano rinunciato ad autonome forme di presenza istituzionale comunale.

La seduta è tolta